La votazione, a scrutinio segreto, avrà luogo per schede, secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 1, del Regolamento.

ai fini della compilazione delle schede, di indicare anche il nome di battesimo dei candidati nell'eventualità di casi di omonimia. Dichiaro aperta

Sospendo la seduta per cinque minuti, che riprenderà con il ricordo della giornata del 25 aprile da parte del presidente Schifani. *(La seduta, sospesa

Onorevoli colleghi, ricorre tra due giorni il 64° anniversario del 25 aprile. Consentitemi di innovare la tradizione della nostra Assemblea che non ha mai visto un dibattito ampio e completo in quest'Aula su una data fondamentale della nostra Repubblica. Ho tuttavia deciso di cambiare questa prassi in quanto ritengo che dopo tanti anni sia finalmente possibile nelle Aule parlamentari riconoscerci in un giorno che deve rappresentare un momento di vera unità per tutti i cittadini. Senza appropriazioni, senza esclusioni, senza spirito di parte, ma invece con una ispirazione che sappia unire tutti gli italiani. Una ricorrenza, quella del 25 aprile, che pur condivisa dalla stragrande maggioranza degli italiani, non è sempre stata di tutti. Credo che i tempi ormai siano maturi perché lo diventi. Il 25 aprile, infatti, costituisce un vero patrimonio collettivo della Nazione perché rappresenta il prezzo pagato da tanti nostri connazionali per la democrazia e la libertà. Dopodomani mi recherò, unitamente al Capo dello Stato e alle altre cariche istituzionali, a deporre una corona all'Altare della Patria. Sarà quello il momento più alto di una giornata che vedrà uniti nel ricordo italiani di tante e diverse generazioni. A cominciare da quella di coloro che vissero in prima persona quegli anni dolorosi e drammatici, ma pieni anche di speranza nel riscatto della nostra Patria e in un futuro di libertà e democrazia. Le ferite, le divisioni, le lacerazioni di quegli anni sono state in grandissima parte superate. E possiamo dire con serenità che questa data vede oggi insieme la stragrande maggioranza degli italiani, uniti - pur nella distinzione chiara delle diverse posizioni - nella memoria e nel ricordo di tutte le vittime. Vincitori e vinti; uomini che combatterono fino al sacrificio; giovani vite spezzate da un odio che attraversò e lacerò le stesse famiglie; crudeltà ed eccidi che si protrassero, purtroppo, anche oltre la conclusione dell'ultimo conflitto mondiale. La ricerca storiografica si è a poco a poco sostituita alla passione politica e la memoria di coloro che combatterono e si sacrificarono per la libertà contro la dittatura fascista viene così mantenuta e trasmessa alle giovani generazioni. Ma vi è anche un sentimento di umana pietà per tutti coloro che, indistintamente, in quegli anni soffrirono e persero la propria vita. È questo forse il frutto più prezioso che dobbiamo conservare: trasmettere alle nuove generazioni - fortunatamente sempre più lontane nel tempo da quegli anni dolorosi - quel messaggio di coraggio, di resistenza all'oppressione, di speranza che tanti giovani di allora vollero mandare. Un conflitto, che aveva visto anche italiani contro italiani, si concludeva in quelle giornate con un'appassionata partecipazione popolare che fu, non dimentichiamolo, parte essenziale delle fondamenta su cui due anni dopo venne edificata la nostra Costituzione. Una Carta che si conserva validamente anche grazie alla lungimiranza, allo spirito di identità nazionale, al superamento dell'odio più acceso con cui uomini saggi di quella generazione - di diverse parti politiche - seppero confrontarsi, garantendo così la democrazia. E che assicura il mantenimento del sacrosanto diritto di libertà conquistato con grande sacrificio anche grazie alla guerra di liberazione suggellata il 25 aprile. È mio augurio che la ricorrenza del 25 aprile, che cade quest'anno in un momento drammatico della nostra vita nazionale che vede migliaia di concittadini colpiti da un terremoto devastante, contribuisca ancora una volta a rinsaldare il vincolo e il patto fra noi italiani. Le forze politiche di maggioranza e di opposizione hanno saputo trovare in questi giorni uno "spirito della ricostruzione" che, lasciando inalterate le rispettive identità, ha saputo cogliere con immediatezza quanto tutti gli italiani - non solo quelli colpiti dal terremoto - richiedevano con forza: un impegno forte, continuo, unitario, non solo dello Stato e delle istituzioni, ma di tutti i partiti e movimenti politici. Spero che questo spirito di unità e di solidarietà possa caratterizzare anche la fase politica che si apre davanti a noi e che il confronto, leale e costruttivo, non cada più nella logica della demonizzazione e dell'aggressione dell'avversario politico. Mi auguro che sappia trovare invece nella ormai non più rinviabile riforma delle istituzioni il suo naturale terreno di incontro. Una Nazione che ha saputo uscire a testa alta dalla tragedia della Seconda guerra mondiale, riconquistando la propria fierezza e il proprio orgoglio, che ha saputo ricostruire dalle macerie un Paese moderno, che ha saputo superare con spirito unitario gli anni bui del terrorismo, che sta oggi affrontando i problemi nuovi posti dalle sfide dell'immigrazione e da una crisi economica globale. Una Nazione che saprà trovare anche in questa difficile occasione quel coraggio, quella solidarietà, quella fiducia nel futuro che il 25 aprile lascia come insegnamento a tutti noi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la celebrazione del 25 aprile 1945, giornata della liberazione nazionale, non ha un carattere rituale. Non è stato rituale il suo intervento, signor Presidente, e non è rituale il dibattito politico, perché quella data è iscritta in modo rigoroso ed impegnativo nella coscienza nazionale, ed è ancora oggetto di riflessioni e di posizioni non sempre condivise. È stato anche opportuno che la storiografia abbia preso il posto di una certa passione politica che degenerava in faziosità per consentire un processo di identificazione di tutta la comunità nazionale attorno a questa data.

saluto ed un ringraziamento a chi ha vissuto quelle giornate, un pensiero grato a chi si è sacrificato per la Patria, per la nostra Nazione, perché quella è stata una pagina straordinariamente incisiva nel percorso di costruzione della nostra identità nazionale e del nostro sentirci comunità. Per questo occorre capire e non soltanto ricordare o celebrare in modo vuoto. Nel nostro Paese ci fu una dittatura, il fascismo, che non fu un evento estraneo al popolo italiano, imposto da forze straniere o da una ristretta classe dominante, ma un fenomeno interno alla Nazione che acquisì un grande consenso di massa, condiviso e radicato in tutte le fasce sociali, popolari e borghesi. Contro la dittatura fascista vi fu una limitata resistenza iniziale, elitaria sul piano culturale e politico. Soltanto successivamente, nell'epilogo drammatico della seconda guerra mondiale e anche in coincidenza con l'occupazione straniera, si scatenò una rivolta morale e armata di larga parte del popolo italiano, che noi definiamo Resistenza. È stato in quella stagione, in quel momento, l'elemento di liberazione nazionale si è mischiato alla contesa politica, al conflitto sui valori politici politici che venivano ad affermarsi; in questa duplicità

alla nostra comunità, a chi in quei giorni si schierò e combatté per la libertà e la democrazia, non posso non ricordare, perché fu parte importante di quel processo, il contributo delle forze anglo-americane, degli alleati: senza quelle forze non sarebbe stata probabilmente possibile la nostra liberazione nazionale. Quella presenza determinante evitò che la Resistenza, la guerra di liberazione si trasformasse in guerra civile, perché è stato a lungo sottaciuto, ma è un dato acquisito, era nella motivazione di alcune di quelle parti in campo la volontà che attraverso la guerra di liberazione si potesse insediare nel nostro Paese un regime politico non democratico.

di tutti, se consapevolmente acquisite, non devono più separarci, ma devono invece far condividere i valori pregnanti e prevalenti di quella fase. Colleghi, senza libertà non può esservi democrazia; senza la libertà tutto è perduto, come amava ripetere il presidente Sandro Pertini. Questo è l'insegnamento che dobbiamo dobbiamo sempre far prevalere. In quegli anni molti uomini e molte donne pagarono con la vita; molti intellettuali che provenivano da tradizioni culturali e politiche diverse furono emarginati, furono confinati e incarcerati. Ma con il contributo di quelle esperienze culturali, immediatamente dopo, abbiamo scritto la nostra Costituzione, attraverso culture politiche che sono quelle che oggi ancora ispirano la vita politica motivo, per tener viva la memoria, ricordare la verità è cosa diversa dalla faziosa rivendicazione di chi vuole ad ogni costo tenersi aggrappato alle proprie posizioni; alle proprie posizioni; la verità del torto e della ragione tra chi combatteva per imporre all'Italia e all'Europa la disumana dittatura nazifascista, la repressione di ogni libertà, lo sterminio dei sottouomini, gli ebrei, gli zingari e gli omosessuali, e chi combatteva sul fronte opposto per realizzare ciò che poi, vincitore, realizzò: la democrazia per tutti, anche per i vinti di allora; la libertà e l'eguaglianza per tutti, senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, com'è proclamato in questa nostra bellissima, moderna, avanzata Costituzione. Viva la Costituzione italiana! Signor Presidente, colleghi senatori, noi vogliamo ringraziarla - e lo facciamo sinceramente - per aver deciso di celebrare in quest'Aula la ricorrenza del 25 aprile. È un atto nuovo e opportuno, che può concorrere a rompere un tabù esistente da troppo tempo su questa ricorrenza, ricorrenza da condividere, che viceversa è ancora oggetto di aspre polemiche politiche. Da queste bisogna sottrarsi una volta per tutte, perché il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani e racconta il riscatto di un popolo di fronte all'oppressione nazifascista, di tutta l'Italia e non solo di una parte. La Resistenza e la lotta antifascista hanno visto in Italia l'impegno condiviso di molti ed opposti orientamenti politici. Cattolici, comunisti, anarchici, liberali, socialisti, azionisti si unirono per combattere le dittature e gettare le basi per la nascita della Repubblica. Nella lotta per la libertà e la democrazia l'Italia della Resistenza pagò un tributo altissimo. Parliamo di circa 45.000 italiani morti, 40.000 tra partigiani e soldati dell'esercito regolare, molte donne. Senza dimenticare che furono circa 40.000 i civili deportati in quegli anni, prevalentemente per motivi politici e razziali, e di questi ne sarebbero poi tornati a casa solo 4.000. Sono tanti gli episodi di eroismo di singole persone come di gruppi partigiani, che in quegli anni di deportazioni, fucilazioni e rappresaglie costituiscono un consolidato, tragico, spaccato della storia del nostro Paese. Questa celebrazione, signor Presidente, ha però assunto negli anni eccessivi contorni politici, nel maldestro tentativo di renderla una ricorrenza di parte. Nessuno può godere di esclusive sul 25 aprile. Questa data non può essere tirata per la giacca da qualcuno che la utilizza come bandiera per estremizzare lo scontro politico. Un siffatto modo di operare ha consentito, in passato, che i nostalgici e i neofascisti trovassero nei ragazzi di Salò l'unica alternativa possibile, contrapponendoli alla Resistenza, come si trattasse di un'altra Italia, di un altro Paese. Si sono messi, insomma, italiani contro altri italiani, colpevoli di aver fatto la scelta sbagliata e di essersi schierati con la Repubblica sociale e con il nazismo. Anche oggi, signor Presidente, questa contrapposizione sembra in alcuni casi tutt'altro che sopita. Assistiamo, da una parte e dall'altra, a rigurgiti estremistici e non di rado violenti. È di pochi giorni fa l'indegna conferenza neonazista a Milano, che ha unito tutti i nuovi estremisti di destra, adoratori di Hitler e negazionisti dell'Olocausto, in una città medaglia d'oro della Resistenza. Così come è grave quell'estremismo di sinistra che brucia le bandiere di Israele in piazza e che accampa pure pretese sulla Resistenza. Oggi, colleghi senatori, il clima del nostro Paese è, per fortuna, tutt'altro rispetto a quello della guerra. Questo ci consente di ragionare sulle colpe, sulle responsabilità di quegli anni, ma non ci ha ancora dato la maturità per affrontare una ricorrenza del genere con la necessaria lucidità, imparzialità e distacco. Per noi la Resistenza rappresenta il no, forte e deciso, che il nostro Paese seppe opporre all'odio nazista, al razzismo, alle farneticanti teorie sulla razza postulate da Hitler. È la base della nostra Repubblica e della nostra Costituzione, è la vittoria della libertà contro l'oppressione, della democrazia sulla dittatura. Sappiamo che probabilmente il presidente Berlusconi sarà con noi ad Onna, la città distrutta dal sisma in Abruzzo, che negli anni della Resistenza subì una dura rappresaglia da parte dei nazifascisti in fuga. Ne siamo contenti, perché è proprio da quel recuperato clima di unità e coesione politica istituzionale e sociale determinato dal terremoto in Abruzzo che possiamo ripartire per intraprendere tutti insieme un percorso di condivisione di momenti, date ed episodi che appartengono alla nostra storia e che devono unire. Non serve dividerci, oltre che, quotidianamente, su tutto o quasi, come impone la politica, anche su date come il 25 aprile, perché questo è davvero un momento di autentico orgoglio italiano. Oggi, cari colleghi, abbiamo una grande occasione: smetterla di litigare sulla nostra storia, inchinarci di fronte ai tanti sacrifici italiani di quella guerra, ai deportati, agli atti di eroismo e ricordare un passo fondamentale verso quella Repubblica che oggi rappresentiamo da questi banchi. Il 25 aprile, il 2 giugno, il giorno del ricordo della Shoah, quello delle foibe, sono legati da un unico comune denominatore: l'indispensabile promozione della dignità della persona umana. Signor Presidente, in conclusione, siamo convinti che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, abbia totalmente ragione. I valori dell'antifascismo e della Resistenza non restarono mai chiusi in una semplice logica di rifiuto e di contrasto. Sprigionarono sempre impulsi positivi e propositivi e poterono perciò tradursi, con la Costituzione, in princìpi e in diritti condivisibili anche da quanti fossero estranei all'antifascismo e alla Resistenza. Perciò il 25 aprile non è una festa di una parte sola. Ecco, dobbiamo festeggiare il 25 aprile con questo spirito. Uno spirito vecchio, perché intriso dei nostri valori repubblicani e costituzionali. Uno spirito nuovo che sa trovare nella nostra Repubblica e nella nostra Costituzione spunti nuovi e attuali per governare e cambiare il Paese.

le parole della "preghiera del ribelle" di Teresio Olivelli, figura esemplare della Resistenza italiana. È cosi che oggi, a nome del Gruppo Italia dei Valori, mi piace fare memoria del 25 aprile. ci troviamo qui oggi per ricordare, a noi stessi innanzi tutto, ma anche ai giovani, al nostro futuro, cosa è stata la Resistenza: un moto di popolo contro l'oppressione fascista e nazista, una volontà seminata tra la gente, che ha dato vita alla nostra democrazia. È stato il sacrificio di una intera generazione che ha combattuto a viso aperto, sulle montagne, nelle vallate, nelle strade, nelle piazze; una generazione fatta di adulti e di ragazzi che provenivano da classi sociali diverse, con idee e ideali di società diversi, uniti da una comune aspirazione: ridare dignità al popolo italiano, risollevare le sorti di un Paese, aprire le porte alla speranza. Viviamo oggi in una società caratterizzata da profonde contraddizioni: da una parte l'esaltazione della conoscenza scientifica quale unica forma di razionalità, dall'altra la tentazione crescente di egoismo e di razzismo. È da poco iniziato il terzo millennio e ancora l'uomo non ha saputo trarre insegnamento dal suo passato; ancora appaiono all'orizzonte bagliori di guerra anche non troppo lontani. Ecco l'attualità della Resistenza: fermarci a riflettere e a cogliere il senso pieno del valore della libertà, valore sacro consegnato alla storia dell'umanità. Sì, sono passati 64 anni dall'aprile 1945. Non sono pochi, e questa Repubblica e questa Costituzione stanno ad attestare in modo inequivocabile l'eredità di quei giorni. il lavoro di autenticazione della democrazia ricomincia ogni giorno e non ammette delega; c'è sempre un rischio per la libertà, dunque c'è sempre il dovere di riconquistarla. Eppure, senza la nostra storia non può esserci memoria di futuro. Allora il mio pensiero va a quei giorni, dove molti furono coloro che presero la via della montagna, soprattutto giovani. Oggi, rileggendo alcune delle loro lettere, si scopre che le loro ultime parole non furono mai di disperazione e di odio ma di speranza e di perdono. Altissimo è stato il contributo in vite umane dato alla guerra di liberazione, nei campi di concentramento e di sterminio, nel corpo italiano di liberazione, con le formazioni partigiane all'estero, nell'isola di Cefalonia e nelle carceri. Il 25 aprile ha visto la resistenza attiva di chi prese le armi come i partigiani e i militari, che seguirono l'impulso della propria coscienza; la resistenza silenziosa della gente comune, dei cittadini che aiutarono e soccorsero i feriti esponendosi a rischi elevati; la resistenza dei prigionieri nei campi di concentramento e di chi rifiutò di collaborare. Oggi, cari colleghi, siamo chiamati tutti ad un nuovo impegno: rafforzare il senso della solidarietà e del comune destino di ogni uomo di fronte alle sfide, anche tragiche, della contemporaneità. Così fecero i partigiani quando imbracciarono le armi animati dal desiderio di sconfiggere il nemico, sì, ma di costruire le fondamenta di una nuova casa comune, di un nuovo modo di vivere e stare insieme. Siamo chiamati, oggi più che mai, come uomini e come cittadini del mondo, ad una rinnovata responsabilità dì fronte a tutta l'umanità. Dobbiamo rispondere con il coraggio dei "ribelli per amore" alle sfide dell'oggi: l'omologazione passiva, l'inconsistenza dei valori, la povertà materiale del Sud del mondo. E allora che dire ai giovani (che sono contento di vedere presenti in Aula), ai giovani di tutte le età? età? Che da quest'Aula, luogo simbolo di un'Italia libera e democratica, si alzi anche per loro un monito: sappiano essere responsabili del loro futuro, coniugando le loro ansie e le loro legittime aspirazioni all'interno di una corretta dialettica democratica. Se sarà così, Se sarà così, il 25 aprile rappresenterà davvero il secondo Risorgimento italiano, una nuova palestra di vita per le generazioni a venire, la difesa dei valori contenuti nella nostra Costituzione, così come ribadito ieri dal nostro presidente della Repubblica, onorevole Giorgio Napolitano: valori di democrazia, di solidarietà, di partecipazione, evitando ogni forma di autoritarismo, per mantenere centrali le prerogative del Parlamento, vero e unico baluardo di libertà. VACCARI *(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopodomani, 25 aprile, ricorre il 64° anniversario della Liberazione dall'occupazione nazista e termine della seconda guerra mondiale, sciagurata e disumana, e noi ci accostiamo con lo spirito di chi sa che ci riferiamo a un momento nodale della storia italiana che va ricordato per il suo significato storico, che andrebbe rinverdito e condiviso per i suoi valori, che solo così possono essere ancora attuali. Libertà e democrazia sono concetti che oggi, specialmente i più giovani, danno per acquisiti. Termini ormai scontati, come se non ci fossero persone che hanno perduto la vita per affermare la nostra libertà e la nostra democrazia. Come inciso, per i veneti come me il 25 aprile è anche un'altra ricorrenza. Cade infatti il giorno del Santo patrono Marco, le cui reliquie, che si trovavano in terra islamica, ad Alessandria d'Egitto, furono avventurosamente traslate a Venezia nell'anno 828 da due leggendari mercanti veneziani: Buono da Malamocco e Rustico da Torcello. Oggi attraversiamo un periodo non facile in una società sempre più complessa, con questioni essenziali ancora irrisolte e che sono diventate più urgenti per la crisi finanziaria internazionale. Credo quindi che sia opportuno riflettere sul futuro del nostro Paese e della nostra comunità.

L'8 settembre 1943 venne meno, e certo non per mancanza di valore, il concetto di memoria storica condivisa, come un ponte crollato tra le diverse ideologie positive. Da allora l'Italia non ebbe più una memoria storica condivisa. A quel ponte crollato, per proseguire nella metafora, si tentò di sostituirne un altro: quello simbolicamente rappresentato dal 25 aprile, quale festa della liberazione dalla dittatura fascista e dall'occupazione militare nazionalsocialista. Dopo di che, però, l'Italia si ritrovò subito divisa in un prima (l'Italia prefascista), in un durante da cancellare (l'Italia fascista) e in un dopo (l'Italia repubblicana e antifascista). Per alcuni la vera Italia rimaneva quella tra le due guerre, per altri la storia d'Italia iniziava dal 1945. Per alcuni la guerra era stata perduta, per altri la guerra era stata vinta. In realtà, tra le due memorie collettive non vi sarebbe più stato alcun ponte. Come non vi sarebbe più stato tra la storia dell'Italia liberale, prefascista, (perché poco apprezzata nella sua integralità, da entrambe le parti) e quella dell'Italia Repubblicana. La memoria condivisa, ovviamente, non può certo essere realizzata con l'amputazione del ricordo della lotta antifascista e della resistenza militare e civile al nazismo del Terzo Reich, ricordo che va invece ripreso, ma in modo non di parte e bandiera di alcuni. Non vogliamo neppure aprire e seguire il percorso del revisionismo e dell'uso della storia e della memoria in funzione *tout-court* di lotta politica. Il punto fondamentale riguarda i civili coinvolti nella resa dei conti, vittime di odi, di ondate di cieca violenza, di meschine vendette personali, esiti tragici e traumatici della guerra civile, che aggiunge quel più di violenza alla barbarie e all'imbarbarimento provocato dalla guerra. Eccidi, violenze, esecuzioni capitali ci furono e ci furono anche a distanza di tempo dalla fine del conflitto ci furono anche deviazioni di frange di area. Occorre anche ricordare gli episodi degli anni successivi alla liberazione, lo sdegno per la mancata punizione di responsabili dei peggiori crimini, l'amarezza per il fallimento dell'epurazione, l'accanimento con cui condanne e arresti fioccarono sugli ex partigiani. È solo l'attenta e meditata contestualizzazione storica che può aiutarci a capire meglio fenomeni tanto tragici e incresciosi, che ancora possono avere riflessi sul nostro presente. La categoria di guerra civile, che pure è stata abnormemente e frettolosamente dilatata in certi studi recenti, andrebbe dimensionata e inquadrata nella vicenda storica del Novecento, se l'obiettivo è quello di apportare un contributo di conoscenza. Urgente ora è la necessità di riformare il Paese, di renderlo moderno e in grado di reggere il confronto e la competizione con gli altri Paesi. Se è vero che il nostro Paese è una democrazia incompiuta, anche questo è uno dei progetti sui quali occorre lavorare per dar vita ad una strategia di riforme, anche costituzionali, che non sia prigioniera delle maggioranze che si alternano. Chiamiamo le giovani generazioni a far vivere e a trasmettere gli ideali sempre attuali di democrazia economica, sociale e culturale. Della Carta costituzionale oggi voglio ribadire i princìpi fondamentali ed insieme i valori legati alle nostre radici cristiane e ricordare come spesso siano invece disattesi. Questo Parlamento ha avuto dai cittadini un mandato speciale: riformare il Paese, non possiamo mancare l'obiettivo e già la prima riforma, il federalismo fiscale, si sta concretizzando. C'è tra l'altro da recuperare il valore morale che viene dal 25 aprile e da quella lotta di liberazione che ha aperto le vie della democrazia e della libertà e ci ha fatto vivere in un Paese che è saputo uscire dalla dittatura fascista, passare attraverso la ricostruzione, svilupparsi, crescere e progredire, diventando un punto di riferimento nello scenario mondiale. Ma non si può vivere di ricordi e non basta evocare il passato perché è facile sfociare in un declino che farebbe scivolare l'Italia in condizioni di precarietà. Il nazismo è stato vinto grazie al sacrificio di donne e di uomini e di nazioni unite contro la barbarie. Ma la minaccia di totalitarismi e terrorismi - di ogni tipo - non è del tutto scomparsa, anzi, la nostra attenzione contro l'ingiustizia e la prevaricazione deve essere sempre intatta. Per queste ragioni, ed in modo propedeutico, il nostro impegno politico deve essere quello di garantire la convivenza civile delle nostre città e non è un caso che il tema della sicurezza sia diventato prioritario in ogni parte del Paese; se non si vive con serenità e in un clima nel quale le libertà individuali siano garantite, i discorsi sulla libertà e sulla democrazia, nel significato solenne che oggi rinnoviamo con convinzione, risultano assolutamente retorici. Anche su questo argomento da subito abbiamo operato in modo fattivo e concreto con approvazioni di provvedimenti anche proprio questa settimana e su questo percorso di fatti continueremo. Noi chiamiamo a rendere attuale la Liberazione, non a vantaggio di cause di parte o strumentalizzando a vantaggio di giuochi di potere, ma per proporre alle generazioni che ci seguiranno di compiere gesti umanitari e profondamente politici nel senso autentico del termine.

Ecco, in queste poche parole vi è il significato del 25 aprile: restituire agli italiani la dignità e il diritto alla libertà. aprile, infatti, non solo rappresenta il ricordo e la commemorazione di tutte le donne e gli uomini che con coraggio e valore restituirono al Paese la speranza di una vita libera dal nazifascismo, ma soprattutto la festa della Liberazione è il vincolo, il patto tra cittadini, il patto di solidarietà, libertà e diritti uniti dal desiderio per un futuro migliore. Il 25 aprile fu uno storico punto di partenza, premessa essenziale per la costruzione di un Paese finalmente democratico, le cui fondamenta sarebbero state poste un anno dopo dai lavori dell'Assemblea Costituente e dal *referendum* attraverso il quale per la prima volta tutti i cittadini - le donne per la prima volta nel nostro Paese avrebbero deciso sovranamente il successivo assetto istituzionale. Valori che aprirono una nuova prospettiva di vita degli italiani e che permisero la ricostruzione economica e sociale del Paese, garantendo a tutti la piena partecipazione politica, al di là delle divisioni ideologiche e politiche che pure erano forti sullo sfondo dello scenario internazionale. Fu questo grande atto di capacità di guardare al futuro che permise all'Italia di avere un ruolo da protagonista nei decenni successivi e di partecipare alla nascita del progetto di una nuova Europa che, in un lento ma inesorabile processo, ha portato a quel bene prezioso rappresentato oggi dall'Unione europea. In un certo senso fu un desiderio di riscattare di fronte al mondo le proprie radici culturali liberali e tolleranti, umiliate dagli anni bui del fascismo, per recuperare un ruolo nella comunità occidentale, e di farsi partecipe di una grande impresa di pace e di collaborazione nel cuore dell'Europa. Oggi, dopo 64 anni il mondo è profondamente cambiato. Tuttavia, non hanno perso validità e attualità le grandi motivazioni ideali della Resistenza e tutte le esperienze attraverso le quali l'Italia seppe rialzarsi dal crollo dell'8 settembre 1943 e farsi protagonista del suo stesso riscatto, della sua stessa liberazione. voglio però aggiungere un passaggio che ritengo importante. Spesso negli anni passati la celebrazione del 25 aprile è stata caratterizzata non tanto dalla gestione di una memoria comune che ebbe valore di fondamento, ma piuttosto da differenze nelle diverse culture politiche, che tendevano a farne un terreno di consenso nelle differenti stratificazioni del tessuto sociale. giunti al 2009, sia necessario, proprio perché ci troviamo di fronte ad una crisi economica internazionale di proporzioni non ancora immaginabili, ad un Paese spaventato, a mutamenti socio culturali di cui forse neanche ci rendiamo conto fino in fondo, assumere la festa della Liberazione come la festa di tutti noi italiani. Dopo il 25 aprile 1945 l'oggetto principale della politica era il tema della guerra e della pace mentre oggi probabilmente è quello della povertà e delle politiche del *welfare*. Due oggetti diversi, ma uniti da una matrice comune: il bisogno di solidarietà tra cittadini e di come riattrezzare il nostro sistema di protezione, di inclusione e di coesione sociale affinché nessuno si senta solo di fronte alle temperie attuali. Oggi come ieri, dunque, la celebrazione di questa festa deve essere non solo omaggio ai caduti, ma simbolico esempio di un vincolo di lealtà e alleanza tra le parti sociali. Riuscimmo allora con questo vincolo ad uscire da una tragedia nazionale. Oggi possiamo insieme riuscire a dare nuove prospettive di sviluppo e nuove speranze al futuro delle giovani generazioni. Riconoscere questa complessità, dare il giusto posto alle diverse tappe e alle molteplici componenti del processo che vide il popolo italiano protagonista del proprio riscatto, non significa rimuovere le distinzioni fra le parti in lotta, né azzerare il passato e cancellare i torti e le ragioni dalla nostra coscienza collettiva. Significa essere davvero eredi di quegli uomini e quelle donne che lottarono e morirono per la nostra libertà: sui monti o nei campi di concentramento, in uniforme o nelle carceri, nascondendo profughi ed ebrei o sfamando sfollati, morendo per fame o sotto tortura. Questa eredità fa del 25 aprile la festa di tutti gli italiani. A tutti coloro che ci hanno restituito un Paese unito, libero e democratico va dunque la nostra profonda riconoscenza e la solenne promessa che non solo non dimenticheremo, ma saremo capaci di storicizzare quei contenuti per avere una Paese migliore e un futuro di pace.

Signor Presidente, colleghi senatori, per parlare del 25 aprile e rispondere all'invito del presidente Napolitano che lo vuole una festa di tutti, è necessario cominciare ponendosi alcune domande: cos'è che ha avuto fine il 25 aprile del 1945? Quanto della realtà storica della Resistenza è entrato nella coscienza civile della Nazione e si è trasformato in senso comune? E quanto invece di un fenomeno così complesso ed articolato che geograficamente ha coinvolto metà dell'Italia e che ha conosciuto diverse manifestazioni è stato sacrificato sull'altare di una narrazione quasi mitopoietica? Ebbene, signor Presidente, crediamo che con uno sforzo di onestà intellettuale da parte di tutti sia possibile ricordare il 25 aprile con la serietà che deriva dalla verità, riconoscendo innanzitutto i grandi meriti degli Alleati ed in particolare degli americani, meriti troppo spesso messi in secondo piano quando non proprio obliterati. E poi, ammettendo che, come ha ben evidenziato uno storico di sinistra, Claudio Pavone, il teatro di quel periodo che oggi va sotto il nome di Resistenza fu, in realtà, il teatro di tre guerre: la guerra patriottica, di liberazione, che portò alla cacciata dei nazisti dal nostro Paese; la guerra civile contro i nazisti e coloro che fino alla fine scelsero di restare fedeli al regime; infine, una vera e propria guerra di classe. noi celebriamo la prima di queste tre guerre, che si lega al senso di Patria che forse l'8 settembre morì, ma che poi è rinato anche grazie al contributo di tanta parte delle Forze armate, nelle quali restò vivo il senso della Nazione. Noi festeggiamo la guerra di liberazione corale, alla quale tutto il popolo italiano prese parte in varie forme. Ma della guerra civile non ci si può dimenticare: della guerra civile tra antifascisti e fascisti, ma anche di quella guerra civile non meno drammatica e profonda che vide contrapporsi agli antifascisti che lottarono contro una dittatura in nome della libertà altri antifascisti, che si batterono in nome di un altro totalitarismo. "Il sangue dei vinti" che ci ha narrato Giampaolo Pansa nasce soprattutto da qui. Infine, signor Presidente, sarebbe bello, e soprattutto sarebbe indice di vera maturità, se nei discorsi di questi giorni non ci dimenticassimo anche di questi altri aspetti che si riconnettono alle nostre celebrazioni e che rappresentano una pagina di storia ancora tutta da scrivere. Ed è proprio la storia che può e deve svolgere una funzione catartica, restituendo unità e serenità al nostro Paese. Signor Presidente, i manuali su cui si sono formate le migliori generazioni di storici - quelli di Renzo De Felice, Rosario Romeo, Gaetano Arfé mettevano in guardia dall'assolutizzazione del concetto di memoria perché spesso - spesso anche in buona fede - la memoria è selettiva, è unilaterale, talvolta persino divisiva laddove di essa se ne fa un cattivo uso politico. Oggi - e questa celebrazione ne è un esempio - vi è la possibilità di restituire alla narrazione della Resistenza la sua complessità, di passare dalla retorica della memoria alla verità della storia, esaltandone la sua funzione catartica. Vi è la possibilità di giungere in nome della verità storica a quella condivisione che sola potrà consentirci di superare il risentimento, di comprendere le vicende ed i comportamenti degli uomini, di chiudere i conti nel senso nobile di questo termine e di andare avanti, recuperando il passato in termini di patrimonio di conoscenza e innalzandoci sopra di esso grazie anche alla potenza del suo insegnamento. *(Applausi

dei fatti che hanno portato a sperare nell'apertura di una fase nuova. Le parole che il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha pronunciato al Vertice delle Americhe l'apertura che è avvenuta in direzione di una nuova fase delle relazioni tra gli Stati Uniti e Cuba prospettano una possibilità che era sembrata molto lontana fino a poche settimane fa. settimane fa. Nella giornata di ieri il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha previsto una crisi abbastanza rapida del regime cubano. Non so se tale previsione sia vera; è certo che le decisioni che saranno assunte a proposito dell'embargo potranno influire profondamente sugli sviluppi della situazione ed accelerare un processo di trasformazione. L'embargo che

data quasi mezzo secolo, può portarci a concludere che mentre l'embargo ha determinato condizioni molto difficili per quanto riguarda la vita dei cittadini del popolo cubano è stato totalmente inefficace nel produrre modificazioni del regime e aperture nella direzione della democrazia. Possiamo dire addirittura il contrario, che che l'embargo è stato utilizzato dal regime cubano, in un Paese nel quale le radici e la cultura patriottiche a partire dalla fine del Ottocento e dall'inizio del Novecento sono così profonde, come un elemento di identità. In fondo, l'embargo ha permesso che il conflitto fosse rappresentato come tra Cuba e Stati Uniti, tra Castro e Bush ultimamente, non come un conflitto essenziale per la democrazia fra il regime cubano ed il suo popolo. Oggi aprire la questione dell'embargo, chiedere al Governo italiano di sostenere una posizione, che peraltro è condivisa sostenuta e riaffermata più volte dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, vuol dire muoversi in questa direzione.

Ne parlo e ne parliamo non per averne letto sui giornali, ma perché questi militanti e questi coraggiosi combattenti per per la democrazia a Cuba li abbiamo conosciuti personalmente. Siamo andati a visitare le loro famiglie quando stavano in galera, abbiamo conosciuto persone che in una situazione difficilissima si sono battute per l'affermazione della democrazia. ha chiesto nei tempi scorsi quanti sono questi oppositori cubani e chi rappresentano. Senza dubbio, è vero che si tratta di una piccola minoranza, ma come si fa a non essere una piccola minoranza in un Paese nel quale

del dissenso cubano credo significhi porre una domanda disonesta. Questa domanda si potrà fare quando le persone saranno libere di esprimersi e quando ci sarà la possibilità di muoversi liberamente, che oggi non è data.

è stata salvata la vita grazie a una mobilitazione internazionale; Vladimiro Roca, che ha passato cinque anni nelle carceri; Elizardo Sánchez, presidente della Commissione diritti umani di Cuba; Oswaldo Paya, che ha rappresentato l'impegno e la mobilitazione di un filone di pensiero cattolico e liberale; Manuel Cuesta Morua, che ha rappresentato l'esperienza socialdemocratica e socialista cubana contro un regime totalitario.

non c'è dubbio, credo che una decisione della comunità internazionale, che il Governo italiano può sostenere, a favore della fine dell'embargo possa accelerare questa prospettiva e questa possibilità.

mandanti di un'azione reazionaria e di rivincita che sarebbe rivolta a restaurare le condizioni di dittatura che esistevano prima della rivoluzione del 1959. Desidero ricordare un dato: i cubani che vivono negli Stati Uniti sono 1.600.000 e i redditi, le rimesse che vengono da questa grande parte della popolazione cubana, sono una delle principali voci del bilancio cubano. Si tratta di una comunità profondamente trasformata nella quale, come in tutti i campi dell'immigrazione, non ci sono più solo i vecchi che ricordano con nostalgia l'epoca di Batista, ma anche i giovani, che chiedono una nuova possibilità di relazione e di rapporto. Pertanto, oggi esistono tutte le condizioni perché, invece che puntare sull'isolamento e sull'embargo, che hanno dimostrato di essere totalmente inefficaci in tutti questi anni, si punti sulla capacità di contagio delle relazioni

dal resto del continente americano. È in nome di questa prospettiva che proponiamo e chiediamo che l'Italia svolga un ruolo effettivo e che si muova perché quelle risoluzioni che per tanti anni si sono ripetute inutilmente all'Assemblea generale dell'ONU diventino oggi operative. Penso che in tutto ciò ci sia qualcosa

di Cuba, infatti, possiamo verificare una politica di intervento attivo del nostro Paese a sostegno dei processi di democratizzazione. Ritengo che in tale contesto si possa fare molto. Alcuni anni fa le ambasciate europee dell'Avana decisero insieme di compiere un atto significativo, invitando alle loro feste nazionali i rappresentanti del dissenso e dell'opposizione.

alla nostra struttura diplomatica in coordinamento con gli altri Paesi europei oggi le possibilità di contribuire ad un'accelerazione dei processi di democratizzazione a Cuba sarebbero molto forti. Questo, in un quadro dell'America Latina che in questi anni ha visto una trasformazione profonda di tutto il panorama: oggi, si tratta di un continente nel quale, a differenza di molti anni fa, la grande maggioranza dei Paesi vive nuove esperienze democratiche e la possibilità della democrazia, in tutto il contenente latinoamericano, non è più solo una speranza.

i progressi realizzati su tanti piani anche nella rivoluzione cubana, solo in questo processo di democratizzazione quegli stessi progressi e quelle stesse conquiste possano essere difesi. della mozione che abbiamo presentato e che chiediamo al Senato di approvare, sperando che il Governo esprima parere favorevole.

Signor Presidente, inizio innanzi tutto rivolgendo un ringraziamento al senatore Marcenaro per aver trovato un'ottima sintesi, tant'è vero che la mozione in esame è stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i Gruppi, poiché tiene conto delle iniziative

i radicali sono stati da sempre vicini ai dissidenti cubani: per anni è stato iscritto al partito radicale transnazionale Francisco Chaviano, che dalle carceri ci informava come poteva,

se è vero che siamo amici di Platone (essendo Platone la bandiera a stelle e strisce), siamo forse più amici della verità: e la verità oggi è che c'è una possibilità di apertura reale, non tanto di dialogo con il regime castrista, quanto se non altro di avvio di un dibattito all'interno della comunità internazionale, che - con atteggiamenti diversi - si è sempre rapportata nei confronti di Cuba, e all'interno del regime castrista stesso. Le dichiarazioni di Raul Castro di apertura o, se non altro, di attenzione e, addirittura, di invito ad un dialogo diretto con Washington su questioni che attengono anche al rispetto dei diritti umani devono essere salutate con soddisfazione

settimana scorsa, poco dopo aver sottoscritto questa mozione, mi sono incontrato con un altro dei dissidenti cubani che vive da una quindicina d'anni in Svezia, il quale mi ha fatto notare il forte rischio che - se non si passa dalla politica sbandierata sui giornali ad un vero e proprio ingaggio sul terreno, inteso come Nazioni Unite, ma anche come rapporti regionali, multilaterali e anche bilaterali con Cuba - il cambiamento di Raul Castro non necessariamente vada verso la libertà

gli atteggiamenti di inerzia diplomatica e recupera una politica che vuole anteporre la ricerca della libertà, e quindi anche la ricerca dalla verità, all'interno di un consesso che invece molto spesso

depositato alcuni mesi fa con la senatrice Poretti - ma addirittura si aumenti perché probabilmente anche dagli intellettuali può venire un ulteriore contributo all'apertura e, finalmente, all'avvio di una transizione verso la democrazia. Infatti, se tale transizione non viene gestita di concerto dalla comunità

per cercare di dare un impulso alla distruzione di un dinosauro politico quale è l'embargo degli Stati Uniti verso Cuba. verso Cuba. Bisogna ricordare anche un altro fatto e cioè che Cuba è forse l'unico Paese dell'America Latina che non abbia avuto una storia di indipendenza: colonia della Spagna fino alla guerra del 1898; in pratica colonia degli Stati Uniti, di fatto giuridicamente, dal 1902 al 1934, dato che il *Platt Amendment* permetteva agli Stati Uniti di intervenire negli affari cubani;

soggetta al duro regime non democratico che tutti noi conosciamo. Dunque, si tratta di mettere fine, ripeto, ad una mostruosità giuridica internazionale come l'embargo su Cuba, che ha avuto varie tappe: è nato all'indomani del tentativo fallito di invasione della Baia dei porci, il 16 aprile del 1961; è stato annunziato da Kennedy praticamente il

senatore Marcenaro ha ricordato che oggi negli Stati Unitici sono 1.600.000 cubani, per i due terzi in Florida, che hanno avuto una grande importanza nel mantenere in piedi la mostruosità giuridica dell'embargo, perché la Florida era lo Stato chiave

cosa sarebbe la Sicilia se il movimento indipendentista del 1945 ed il suo braccio armato avessero vinto i primi confronti armati con i carabinieri, se Antonio Canepa si fosse rifugiato sulle Madonie e qualche servizio segreto straniero avesse in qualche modo fomentato una rivoluzione vittoriosa

e la diaspora siciliana in Italia fosse tagliata dalle sue radici isolane. Poniamoci in queste prospettive storiche.

Invita i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo dei voti.

mozione si chiede al Governo un impegno concreto per dare finalmente attuazione al voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che quest'anno, per la diciottesima volta consecutiva, a larghissima maggioranza ha approvato una risoluzione che chiede la rimozione dell'embargo economico, commerciale e finanziario nei confronti di Cuba. Veniva ricordato in precedenza dai colleghi che è passato ormai mezzo secolo da quando ha avuto inizio l'embargo deciso allora dal presidente Kennedy e tantissima strada si è fatta, molto è cambiato nello scacchiere politico centro-sudamericano. Cuba resta però un'isola in piena crisi, economicamente allo stremo, e dall'embargo quest'isola ha ricavato solo ulteriore povertà, sentimenti populisti, una chiusura ed un'ostilità nei confronti del resto del mondo e del modello occidentale che sono a fondamento dell'oltranzismo politico e degli eccessi del leader storico Fidel Castro. Nel Paese esistono ancora enormi restrizioni accentuate dall'embargo ed è evidente che ci troviamo in un contesto nel quale le libertà fondamentali sono assolutamente vulnerate, a partire dalla libertà d'informazione, e gli abitanti dell'isola sono ovviamente combattuti fra la lealtà a Fidel Castro o al fratello Raul e le molte tentazioni cosiddette capitaliste. Qualche recente apertura di di Raul ha fatto pensare ad un miglioramento della situazione ma, al di là di qualche buona intenzione, purtroppo sembra che stia cambiando troppo poco. Ciò che invece sta avvenendo, ed è importante, è il ricambio generazionale che si sta verificando; sta uscendo dalla scena politica quella vecchia classe legata alla rivoluzione che ha dominato negli ultimi anni e che ora sembra possa essere sostituita da una classe dirigente più matura e aperta al cambiamento e all'evoluzione politica e culturale. Da qui la necessità di superare, con scelte politiche internazionali coraggiose, il patriottismo estremo e il populismo di Castro e del suo *entourage*, che peraltro mostrano evidenti limiti e contraddizioni, posto che l'economia gira a vuoto, la popolazione è allo stremo e le poche conquiste del castrismo non bastano a soddisfare più i crescenti bisogni dei cittadini cubani, i quali tentano di accedere in ogni modo ai mezzi di informazione e ai beni di consumo e ad un diverso stile di vita rispetto a quello proposto dal regime. In altri termini, signor Presidente, posto che l'embargo si è tradotto in un disastro per l'economia cubana, senza che a ciò si sia obiettivamente accompagnato il previsto sovvertimento del regime, anzi, questo negli anni si è consolidato, questo negli anni si è consolidato, credo che una scelta di realismo politico, oltre che doverosa rispetto anche agli scenari che si stanno prefigurando, a cominciare dalla nuova presidenza Obama, ci porti a dover sostenere con maggior vigore e con maggior forza l'iniziativa italiana in sede ONU; per non parlare poi della circostanza che negli Stati Uniti vivono 1.300.000 cubani, le cui rimesse sono il sostegno economico fondamentale, oltre agli emigrati in Messico, Spagna e Portorico, per l'economia reale di quel Paese. Ciò che però è necessario evidenziare conclusivamente è che questa iniziativa deve essere accompagnata da un'iniziativa altrettanto forte che punti non solo all'eliminazione dell'embargo, ma anche alla liberazione dei numerosi detenuti e prigionieri politici in quel Paese Paese e ad un'apertura chiara e netta verso la reale democratizzazione di quel Paese per evitare il rischio di un'altra deriva populista e della possibilità che ad un regime se ne sostituisca nel tempo un altro in ragione di bisogni economici e sociali non soddisfatti dei cittadini cubani. Per queste ragioni, signor Presidente, in maniera convinta ringraziamo il collega Marcenaro e gli altri colleghi firmatari della mozione n. 104 e voteremo a favore della stessa. Siamo compiaciuti anche della circostanza che il Governo abbia espresso parere favorevole.

si intende il blocco degli scambi totale, deciso unilateralmente da un solo Paese nei confronti di un altro Paese e basato su motivi esclusivamente politici. Si tratta, potremmo dire, dell'utilizzo di uno strumento che appare, più che di diplomazia, come un mezzo di guerra, anche se di guerra economica stiamo parlando. È un fatto dimostrato che gli embarghi economici, soprattutto quelli totali, non portano ai risultati che si vorrebbero conseguire. Infatti, la privatizzazione dei beni di prima necessità, dei fondi economici, degli strumenti di sopravvivenza ad una intera popolazione ha come effetto che la popolazione si stringe attorno al Governo in carica, dato che solo da questo può ricevere i mezzi per sopravvivere, e coltiva la cultura dell'odio verso le Nazioni che hanno stabilito l'embargo. Tuttavia, si è fatto largo uso dell'embargo e lo strumento è pericolosamente tornato di moda - permettetemi l'espressione - nell'opera di contrasto al terrorismo. Una normativa statunitense sul commercio estero risalente al 1979 prevede tali sanzioni contro i Paesi periodicamente elencati dal Governo americano nella cosiddetta *terrorist list*, la quale attualmente enumera Iran, Iraq, Libia, Siria, Sudan, Cuba e Corea del Nord. Nord. Il caso di Cuba, rispetto agli altri, rappresenta tuttavia un *unicum* anche per un Paese come gli Stati Uniti, assai avvezzo all'utilizzo dell'embargo. Le prime misure economiche contro Cuba furono prese nel 1960 e gradualmente estese. Nel 1963 l'embargo fu completato. Esso è stato finora costantemente mantenuto con poche varianti. Negli ultimi anni si è anche avuta un'ulteriore *escalation* di tali misure, prima con l'adozione del progetto di legge presentato dal deputato Torricelli, il *Cuban Democracy Act* del 1992, poi con la legge Burton, un provvedimento che inasprisce ulteriormente l'embargo, penalizzando le imprese straniere che hanno affari con Cuba e consentendo a cittadini americani di far causa ad investitori stranieri che utilizzino proprietà espropriate dal Governo cubano. Tuttavia, questa situazione immutata per ben quarant'anni, cari colleghi, sembra si stia sbloccando con una rapidità crescente nelle ultime settimane. Quello che ci chiediamo è se il colosso America e l'intransigente Cuba si stiano veramente avviando verso la fine di questa guerra fredda. Per ciò che riguarda Cuba, è certo che esistono segni che possa davvero arrivare un cambiamento cinquant'anni dopo la rivoluzione che portò Fidel Castro al potere. Con una mossa inaspettata, infatti, Raul Castro, fratello di Fidel, ha recentemente licenziato decine di alti ufficiali, esponenti della linea dura del Governo. È un fatto, questo, che ha segnato il primo anno da presidente di Raul ed ha aperto concrete speranze che Cuba possa andare oltre quelle piccole riforme finora introdotte. Per ciò che riguarda gli Stati Uniti, sempre più cittadini americani e sempre più esponenti politici ritengono che l'embargo economico non abbia funzionato. O meglio, permettetemi di dire, funziona ed ha funzionato per Nazioni come il Canada, la Corea del Sud e dozzine di altri Paesi che hanno fatto e fanno fortuna fornendo a Cuba cibo e materiali per costruzioni. Le critiche all'embargo arrivano anche sulla scorta di motivazioni non solo altruistiche nel considerare i bisogni del popolo straniero: i membri del Congresso americano, che lamentano l'esternalizzazione dei lavori stanno sempre più ponendo all'opinione pubblica il problema che l'embargo su Cuba priva di occupazione migliaia di lavoratori americani. Obama, attenta sia alle aperture multilaterali che ai bisogni dei cittadini americani, sembra quindi giunto il momento per Washington di agire. Ed i primi passi mossi dal presidente americano in questo senso sono più che positivi: è dei giorni scorsi, infatti, la decisione che permette ai cubano-americani di spedire soldi ai parenti a Cuba e di visitarli regolarmente, con l'attenuazione anche delle restrizioni ai viaggi per tutti gli altri. colleghi, la fine dell'embargo non è immediata - questo è un fatto tangibile - e anche se bisognerà ancora aspettare, tuttavia i buoni auspici ad oggi ci sono. Premesso tutto ciò, vorrei dire che la mozione che ci accingiamo a votare oggi costituisce l'ennesimo tassello, l'ulteriore spinta propulsiva per realizzare davvero la fine dell'embargo, ed il suo valore aumenta proprio perché la situazione internazionale nuova, degli ultimi mesi, degli ultimi giorni, ha reso probabile ciò che prima appariva, ad essere ottimisti, solo lontanamente possibile.

si chiede al nostro Governo di agire in tutte le sedi possibili per il superamento dell'embargo. Sarebbe un grande risultato se, già durante l'appuntamento internazionale che ci vede maggiormente coinvolti, il G8, si arrivasse ad avere qualche certezza maggiore sulla fine del blocco economico. Certo, come affermato dallo stesso Presidente americano, gli USA restano in attesa di decisioni concrete da parte dell'Avana, e tali passi dovrebbero essere mossi fondamentalmente nel campo della tutela dei diritti dell'uomo. Dunque, ritengo importante che nella mozione sia stato inserito l'invito al Governo a chiedere alle autorità cubane la liberazione dei prigionieri politici detenuti nelle loro carceri. carceri. Cari colleghi, è vero che gli USA sono il Paese più potente e ricco del mondo, ma è anche vero che sono un solo Paese e che i problemi che affrontano non possono essere risolti da un unico Paese. Mi viene da dire che, laddove le armi hanno fallito (si pensi all'Afghanistan o all'Iraq), potrà di più l'economia e il fascino esercitato dal modello di sviluppo occidentale, in quanto questi pongono, come moneta di scambio per la democratizzazione, beni e servizi appetibili per la popolazione cubana. Dunque, concludendo, signor Presidente, annunci il voto positivo del Gruppo dell'Italia dei Valori alla mozione che è sostenuta da tutte le forze politiche per la fine dell'embargo cubano. L'Italia dei Valori crede fortemente nella possibilità che il processo di democratizzazione abbracci ogni Paese, ed auspica che, a vent'anni dalla caduta del muro di Berlino, segua la caduta di questo ultimo muro residuato dalla Guerra fredda, fatto di limitazioni economiche che hanno soffocato e soffocano le persone. Pertanto, anche a seguito delle prime avvisaglie di apertura date da entrambi i Governi, quello cubano e quello statunitense, davvero mi auguro che questa positiva rivoluzione nelle relazioni fra i due Paesi sia possibile, e che lo sia anche grazie al contributo italiano sintetizzato in questa mozione che è, come dicevo, *bipartisan*, quindi a maggior ragione

colpisce quindi interessi di singoli privati americani e grosse compagnie americane creando una riforma irreversibile, ponendo dei paletti: si proibiva la successiva vendita dei terreni, l'affitto o il frazionamento delle nuove unità. Castro continua nella sua azione e nel 1960 nazionalizza tutte le compagnie petrolifere dell'isola, prevalentemente compagnie americane, la Standard Oil, la Texaco, la Esso, e anche una britannica, la Shell; quel provvedimento venne firmato dall'allora ministro dell'industria, che rispondeva al nome di Ernesto Che Guevara. Gli americani non possono non far nulla

e i medicinali. Castro - a questo punto, è una guerra fredda - chiede che venga ridotto completamente il personale residuo dell'ambasciata USA a L'Avana. L'America percepisce; siamo nell'epoca della guerra fredda, dei grandi blocchi. Sappiamo che Kennedy non era un guerrafondaio, probabilmente, faceva parte della visione politica che tanta sinistra oggi richiama in quest'Aula, però sentì il dovere di provare a sovvertire l'ordine e il regime castrista: ahimè, un grande fallimento. Tutti ricordiamo l'esito dello sbarco nella Baia dei

un aiuto all'allora URSS; si allacciano subito rapporti commerciali, i russi chiedono di poter acquistare tutte le partite di zucchero invenduto, in cambio di partite di petrolio, però pretendono l'installazione di missili sovietici sull'isola. Prende avvio così una grande operazione diplomatica e Kennedy riesce sostanzialmente a depotenziare questo pericolo di *escalation*, effettivamente, a questo punto, armata, e non più embargo commerciale; in cambio si negozia lo smantellamento di tutte le basi missilistiche americane allora presenti in Turchia.

tutte le precedenti restrizioni per i viaggi americani verso Cuba e le rimesse dei cubani americani verso il Paese d'origine. l'operazione di Obama tende a rendere meno dipendente il popolo cubano dal regime di Castro. Veniamo ora alla nostra azione.

È un po' come la crisi Italia-Libia: dopo settant'anni abbiamo risolto il problema dei danni di guerra il cui ristoro ogni giorno la Libia chiedeva al nostro Paese.

tocca soltanto gli Stati Uniti d'America? È una questione bilaterale, che sembra si stia distendendo, ma non per interventi esterni; infatti, nemmeno le risoluzioni ONU

sarà sempre auspicabile nei confronti di qualsiasi tipo di regime. Come Lega Nord, avremmo gradito magari un elemento in più in questo documento. Una frasetta sarebbe infatti risultata molto opportuna: ricordare l'aspetto dei diritti umani,

vengono processate in piazza le persone, non vengono celebrati processi sommari, ma vi è una limitazione di democrazia dei diritti, un'invadenza di una polizia che probabilmente non ha eguali. Ci troviamo in una Assemblea, in un emiciclo in un emiciclo politico e capiamo cosa vuol dire non avere la possibilità di protestare o di mettere in piedi un partito perché immediatamente sarebbe non solo sciolto, ma repressi e incarcerati i suoi esponenti, in quanto ogni partito fuori di quello di Governo sarebbe un esempio di nemico contro lo Stato e pertanto da reprimere immediatamente. Due parole su questo si potevano dire senza voler alterare il contenuto di tutto

Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore della mozione. Ringraziamo il Governo per aver espresso parere favorevole. L'occasione della dichiarazione di voto ovviamente

della costituzione della NATO. Le due date ci portano a riflettere su come tanto siano cambiate le cose dal 1962, forse uno degli anni di crisi più acuta nel rapporto fra i due blocchi di allora che portò all'esasperazione massima delle sanzioni nei confronti di Cuba. Ricordare questa data mette in evidenza anche le contraddizioni che il mondo oggi ci propone nelle relazioni multilaterali. Per esempio, una delle ragioni di fondo per cui gli Stati Uniti d'America iniziarono un'azione di pressione negativa nei confronti del regime che si era imposto a Cuba dopo la rivoluzione fu che non era tollerabile avere un Governo comunista alle porte.

assolutamente inconcepibile e, quindi, non per sposare una tesi piuttosto che l'altra, metto in evidenza queste contraddizioni di oggi. Aggiungo ancora che si fa l'embargo nei confronti di Cuba perché è un regime comunista e poi, in realtà, si hanno con la Repubblica cinese rapporti economici che, anzi, vengono portati come esempio per essere rafforzati e rilanciati. Oggi tutti siamo d'accordo che

G20. Questi elementi li richiamo per dire quanto sia anacronistico che l'embargo verso Cuba esista ancora. In realtà, il presidente Obama ha fatto un primo gesto di buon senso. Rendendosi conto che non poteva revocarlo dalla mattina alla sera, ha cominciato a togliere una parte di quegli elementi che rendono questa vicenda assolutamente anacronistica. È chiaro che nella nostra mozione noi sosteniamo che

a Cuba e, quindi, un'affermazione dei princìpi di democrazia che sono stato ricordati e che ancora in questo momento in quella realtà sono venuti meno.

a quante malefatte si sono costruite intorno a questa clausola che l'ONU aveva concesso per ridurre il peso dell'embargo su Poi, in realtà, per risolvere il problema si è dovuto fare una guerra perché l'embargo non aveva prodotto alcun risultato positivo.

vuole essere un attore importante in questa evoluzione dei rapporti multilaterali nel mondo. Pertanto, deve dire una parola chiara sul fatto che l'embargo su Cuba grida vendetta

non esistono. Sono questi gli elementi che dovremmo più liberamente mettere in evidenza, immaginando che la ragion di Stato, che nel passato è stata invocata in tante occasioni, comincia a fare acqua da tutte le parti.

nei luoghi internazionali e concorre a prendere decisioni. In ogni caso è in grado di fare una relazione organica fra ciò che si dice e la prassi di ciò che si fa. Questo è il senso profondo

invitare il Governo a cogliere le novità positive che l'amministrazione americana ha cominciato a rendere evidenti e concrete, passando dalle enunciazioni di campagna elettorale agli atti concreti che man mano si stanno affermando. Un'ultima considerazione

non funziona. Noi non abbiamo mai messo in discussione il nostro rapporto di amicizia, cosa diversa dalla condivisione piena di ciò che l'amministrazione che governa quel Paese fa e pratica; anche quando è stata più aspra la differenza fra noi, nel dibattito interno nazionale, rispetto a quella politica estera, nessuno di noi ha mai messo in discussione la lealtà atlantica e il rapporto di amicizia con gli Stati Uniti. Ma oggi questi ultimi stanno cambiando gradualmente ma concretamente la loro politica estera. Cominciano a manifestare un'altra visione del mondo, mondo, a pensare che i rapporti che si devono realizzare fra i Paesi per governare globalmente il mondo non possono essere impostati o ispirati a quei princìpi ai quali era ispirata la politica verso il mondo dell'amministrazione precedente.

in grado di costruire un'azione futura che sia effettivamente all'altezza del ruolo che giustamente chi rappresenta questo Paese nelle sedi multinazionali vuole esercitare (e tutti insieme dobbiamo sostenere questa linea), è bene ricordare e sottolineare che se l'unità si costruisce sinceramente e su basi solide, queste ultime sono tanto più solide quanto più è chiaro il percorso che diversamente abbiamo attraversato per arrivare all'unità di oggi. *(Applausi

realtà che dà segni di voler anch'essa abbandonare certe posizioni troppo rigide. Mi limiterò a sottolineare tre elementi che, d'altra parte, qualche altro collega ha già sottolineato prima di me. Il primo -

dei prigionieri politici e dei diritti umani in quel Paese, facciamo però la corsa ad avere rapporti economici

e per molti versi perfino controproducente rispetto agli stessi motivi che vengono addotti a giustificazione dell'embargo. Credo che praticamente le misure nei confronti di Cuba in particolare abbiano ampiamente dimostrato non soltanto di essere inefficaci,

della posizione statunitense che il nuovo Presidente sta adottando nei confronti di alcuni Paesi, soprattutto di Cuba. Credo che, a cominciare dalla revisione delle restrizioni applicate alle visite familiari - il collega Marcenaro qualche cosa ha detto a questo proposito - fino al problema dei prigionieri politici, gradualmente il rapporto Stati Uniti-Cuba stia cambiando. E dico agli amici della Lega che non può che essere così, perché una rivoluzione troppo spinta dei rapporti degli Stati Uniti con Cuba non sarebbe nemmeno gradita a Cuba, perché i progressi che questo Paese sta facendo devono essere

concernessero misure concrete che passo per passo, però, portassero quel sollievo, quella liberazione della popolazione, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani,

quella di cominciare a dialogare da parte del mondo occidentale con l'opposizione democratica, che pure esiste a Cuba. Ed è vero quanto è stato ricordato: questa opposizione democratica non possiamo certamente quantificarla, per per ovvi motivi, ma siamo certi (perché chi è stato a Cuba ed ha parlato con i cubani ne ha avuto la precisa sensazione) che non si tratti soltanto di intellettuali o filosofi che immaginano

il 16 ottobre, a Parigi, in un dialogo tra le autorità cubane e la *trojka* dell'Unione europea, il problema della possibilità che vi siano altre opinioni manifestate esteriormente da parte di strati della popolazione non d'accordo con il regime è stato evocato. Quindi, si tratta già di un progresso che stiamo ottenendo. A questo punto, ovviamente, spetta alla Presidenza attuale dell'Unione europea dare continuità a tale dialogo, che non è solo teorico, perché voglio ricordare che nel frattempo la cooperazione allo sviluppo europea ha più volte inviato mezzi finanziari e concreti per l'assistenza alla popolazione cubana colpita dagli uragani tropicali della fine della scorsa estate. Abbiamo quindi già aperto un canale pratico di interventi in aiuto di questa popolazione ed abbiamo aperto un canale politico di dialogo con le autorità cubane per la politica cubana e con l'opposizione, ancora abbastanza sommersa, per fare in modo che la somma di questi tre fattori consenta uno sblocco, ripeto, certamente non in breve tempo, ma, ci auguriamo, anche in tempi non troppo

Presidente, ho chiesto la parola per esprimere la più viva e sincera preoccupazione per le sorti di Eugenio Vagni, l'operatore della Croce Rossa rapito nelle Filippine il 15 gennaio scorso. Queste sono ore di particolare angoscia per i familiari; infatti, proprio dalle prime ore di stamani, seguono notizie discordanti sul destino del proprio congiunto, che ora potrebbe essere nelle mani di un altro gruppo di ribelli. Inizialmente si era pensato infatti che l'operatore fosse stato abbandonato dai suoi rapitori, ma secondo il capo della polizia locale ci sarebbe stato soltanto uno scambio, nonostante le condizioni di salute dell'ostaggio, che non dovrebbero permettere grandi spostamenti; avrebbe problemi di deambulazione. Vagni, lo ricordo anche all'Assemblea, è l'ultimo di tre dipendenti del Comitato internazionale della Croce Rossa, rapiti sull'isola di Jolo il 15 gennaio scorso, da una prigione in cui i tre avevano compiuto un sopralluogo nell'ambito di un progetto di ristrutturazione idrica. Pertanto, Presidente, mi permetto di invitare la Presidenza e, per suo tramite, il presidente Schifani a sollecitare il Governo ad intraprendere le necessarie azioni diplomatiche per avere al più presto notizie sulle condizioni di salute di Eugenio Vagni e richiederne l'immediata liberazione. La ringrazio, senatore Filippi, per il suo intervento. La Presidenza condivide le preoccupazioni da lei espresse per la sorte del nostro connazionale.

Signor Presidente, prendo la parola per ricordare alla Presidenza e all'Aula, alla vigilia del 24 aprile, che domani è celebrata in tutto il mondo la giornata (si tratta del genocidio armeno. Lo ricordo anche a nome dell'Intergruppo parlamentare di amicizia Italia-Armenia, recentemente costituitosi, che vede presenti i parlamentari di tutti i Gruppi politici di Camera e Senato. Domani mattina le comunità armene di Roma ricorderanno la grande sofferenza storica non solo del popolo armeno, ma dell'intera area europea e per le comunità armene della diaspora nel mondo. Questo momento verrà ricordato domani mattina alle 11, nella chiesa degli armeni in via Giulia a Roma, Volevo ricordare questo evento al Parlamento italiano perché la coscienza del genocidio che oggi continua a dividere, ma vede anche momenti di ricerca comune tra i popoli coinvolti nella vicenda - possa avere attenzione e sostegno

ma anche per il dovere che abbiamo, perché un futuro di pace e di convivenza non si costruisce dimenticando le tragedie del passato:

diverrebbe responsabile se quel genocidio non venisse assunto come esistito, come condanna comune e come impegno a guardare oltre. Da questo punto di vista, la pacificazione che c'è stata in Europa rispetto al nazismo si è basata proprio su questo: non dimenticare un'atrocità saper guardare oltre. L'episodio che mi è rimasto sempre in mente - Mitterrand e Kohl che si danno la mano di fronte al cimitero nelle Ardenne - è uno dei momenti su cui dobbiamo e dovremmo costruire anche

Siamo tutti d'accordo che c'è stato un eccidio e che sicuramente tale vicenda è stata strumentalizzata da ambo le parti; affiderei però alla letteratura scientifica,

l'occasione sarebbe quella di evitare di utilizzare tale avvenimento come ulteriore paletto posto di fronte all'ingresso della Turchia nell'Unione europea, perché, allora sì, è certo che non si andrebbe nella direzione auspicata da tutti quanti.

seduta fino alle ore 13, per consentire ai senatori Segretari di completare lo spoglio